Grazie,

È comprensibile il loro atteggiamento, anche se non è giustificabile, viste le condizioni. Chiedo a lei, signor Presidente, come seconda carica dello Stato, di

Quindi, credo che tutti insieme dobbiamo far sentire una voce pacata, ma anche autorevole, nei confronti di una società straniera, come la Yamaha che vuole mantenere la sua attività commerciale in Italia, ma eliminare l'attività produttiva, privando

Signor Presidente, colleghi, la Camera dei deputati ha approvato alcuni emendamenti al disegno di legge di bilancio trasmesso dal Senato. In particolare, tali modifiche si sono rese necessarie ai fini di una migliore allocazione della spesa in seguito all'emanazione dei regolamenti di organizzazione di alcuni Ministeri. Altre modifiche si sono rese necessarie per tener conto dell'istituzione del Ministero della salute, previsto dalla legge 13 novembre 2009, La tabella 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata interamente sostituita al fine di tener conto del regolamento di organizzazione del suddetto Ministero, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 240, che ha modificato l'articolazione delle direzioni generali del Ministero stesso. Per quanto concerne i risultati differenziali di bilancio, come integrati con le modifiche apportate alla legge finanziaria, il saldo netto da finanziare non varia rispetto a quello risultante dopo l'esame dei documenti di bilancio effettuato dal Senato. Esso resta pari a circa 62 miliardi di euro. Il risparmio pubblico passa da 18,981 miliardi a 18,235 miliardi, facendo registrare, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, un lieve miglioramento. Concludendo, signor Presidente, colleghi, dalla valutazione fatta, anche sulla scorta del dibattito svoltosi in Commissione bilancio, in conclusione di questa terza lettura, possiamo dire che, complessivamente, questo bilancio si inscrive in una situazione

anche della condizione di finanza pubblica che abbiamo davanti. Dobbiamo provare tutti a cambiare i fattori di contesto che oggi fanno spesso fuggire, come osservato,

Occorre quindi trovare uno spunto e uno spirito riformatore, magari in un clima di concordia nazionale che sfugga alla tentazione di un bipolarismo distruttivo, che affronti il tema della riduzione e della qualificazione della spesa pubblica. le riforme avviate in questa legislatura vanno in questa direzione: quella del pubblico impiego, il federalismo fiscale, la riforma della scuola e dell'università, la riforma della giustizia civile e da ultimo - ma non per ultima - la riforma della legge di contabilità dello Stato, che dovrebbe assicurare uno sguardo più sistematico e pervasivo sulle spese del comparto pubblico e sulla qualità dell'impiego delle risorse pubbliche. A valle di questo processo riformatore dovremmo ottenere risparmi importanti da destinare alla riduzione selettiva del carico fiscale, come richiesto come richiesto da più parti, a favore delle imprese e delle famiglie che potrebbero aiutare una più spedita ripresa, al fine di raggiungere quei livelli produttivi bruciati in questi anni di crisi globale. Questo, colleghi, è l'auspicio; questo è il compito che abbiamo davanti. Signor Presidente, rispetto al disegno di legge finanziaria licenziato in prima lettura, la Camera dei deputati ha notevolmente incrementato il contenuto della manovra. Infatti, il disegno di legge finanziaria presentato al Senato in terza lettura consta, all'articolo 2, di 243 commi rispetto ai 55 licenziati in prima lettura. Le numerose modifiche apportate, pur determinando una ricomposizione del quadro contabile per via del notevole incremento della sua misura lorda, hanno mantenuto sostanzialmente invariati gli effetti netti sui saldi di finanza pubblica rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato. Tra le modifiche apportate, si segnalano, in particolare, i commi da 5-*bis* a 5-*quater* dell'articolo 2, che riducono di 20 punti percentuali l'acconto IRPEF 2009, prevedendo, per coloro che non hanno applicato la riduzione dell'acconto, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione o, se lavoratori dipendenti, la corresponsione dell'eccedenza negli emolumenti di dicembre. I commi da 56 a 94 danno attuazione al Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Viene incrementato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, mentre per l'anno 2012 si prevede un incremento del 2,8 per cento rispetto al livello di finanziamento relativo all'anno 2011. Inoltre, è rideterminata l'annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, confermando al 97 per cento delle somme spettanti la percentuale ordinaria delle anticipazioni e al 98 per cento quella per le Regioni virtuose. Nel contempo, sono incrementati da 23 a 24 miliardi gli investimenti per l'edilizia sanitaria. Un'apposita disciplina è disposta per le Regioni che non garantiscono l'equilibrio economico sanitario, prevedendo, in caso di mancata attuazione delle misure di rientro, l'incremento automatico delle aliquote fiscali regionali e la decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari. Le Regioni con piani di rientro per l'estinzione dei debiti pregressi fino al 2005 avranno da parte dello Stato un'anticipazione di liquidità pari a un miliardo di euro. Infine, si stanziano 400 milioni per l'anno 2010 sul fondo per le non autosufficienze. I commi da 96 a 115 adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. I commi 117 e 118 dispongono il rimborso ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'ICI sull'abitazione principale, procedendo ad integrare delle dovute risorse lo stanziamento finalizzato allo scopo. I commi da 120 a 150 prevedono poi una serie di misure destinate al sostegno del reddito dei lavoratori, al mantenimento dei posti di lavori o alla riassunzione di disoccupati stabilendo, tra l'altro, anche la proroga per il 2010 della detassazione dei contratti di produttività. Per l'intero "pacchetto quantificata nel triennio 2010-2012 una cifra pari a circa 1,4 miliardi di euro. I commi da 151 a 172 sono diretti ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle Regioni del Mezzogiorno e a sostenere le iniziative imprenditoriali. A tal fine è prevista la costituzione, che non riuscimmo a portare a termine qui in Senato, della Banca del Mezzogiorno spa, partecipata dallo Stato quale socio fondatore e da altri soggetti privati. Tra le misure di razionalizzazione, si segnalano i commi da 173 a 178, che dispongono la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a Comuni e Province e dei contributi spettanti alle comunità montane. A fronte di tale riduzione di risorse, gli enti citati potranno ridurre alcune voci di spesa riducendo il numero dei consiglieri, degli assessori e sopprimendo la figura del difensore civico, la figura del direttore generale e l'istituto dei consorzi di funzioni tra gli enti locali. contenute in altri commi, afferiscono alle spese di giustizia e principalmente alla semplificazione della pubblicazione delle sentenze e alle modifiche del contributo unificato. I risparmi di spesa e le maggiori entrate così realizzate sono destinati alle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria. Sul fronte degli investimenti si introducono ulteriori disposizioni finalizzate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina: in particolare, si autorizza la spesa di 470 milioni per il 2012, quale contributo ad ANAS spa per la sottoscrizione e l'esecuzione di aumenti di capitale della società Stretto di Messina spa. Ancora, il comma 209 stanzia 500 milioni di euro per l'attuazione del programma di edilizia carceraria finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all'aumento della capienza di quelle esistenti. Relativamente agli investimenti destinati alla sicurezza dei cittadini si ricordano il comma 229, recante disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole, e il comma 230, che destina un miliardo di euro per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. del problema della sicurezza, sono strate introdotte alcune norme in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni che prevedono minori restrizioni nelle procedure di assunzioni di personale nei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco nel triennio 2010-2012. Anche il settore della ricerca e dello sviluppo risulta interessato da alcune disposizioni. In particolare, il comma 226 incrementa di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta relativo alle spese in ricerca e sviluppo. Infine, in numerose disposizioni del disegno di legge finanziaria è previsto il trasferimento di risorse al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, ed il contestuale utilizzo delle medesime a copertura finanziaria di interventi specifici. In particolare, allegato al disegno di legge, compare un elenco con una serie di finalizzazioni finanziate, per l'appunto, con le disponibilità del Fondo in questione che residuano agli utilizzi contenuti nell'articolato del disegno di legge. Tra queste si segnalano: si segnalano: il finanziamento della proroga della devoluzione della quota del 5 per mille dell'IRPEF; quello degli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici; l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; il sostegno alle scuole non statali; interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto; la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

a 8,9 miliardi, di cui 3,7 provenienti dallo scudo fiscale e 3,1 dal TFR, con circa 2,1 miliardi di tagli o rimodulazioni; alla fine la spesa vera, però, è di soli 5,2 miliardi. nel corso dell'esame alla Camera sono stati sostanzialmente, e in parte, una risposta anche a richieste che provenivano già dal Senato in prima lettura; in alcuni casi è come se alcuni emendamenti, presentati e respinti da maggioranza e opposizione qui in prima lettura,

l'adeguamento e la messa a norma antisismica, nonché i 400 milioni all'università, gli 854 milioni di credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca, su cui tanti emendamenti e tante richieste soprattutto dall'opposizione. Vi è poi tutto il pacchetto sugli ammortizzatori sociali che, come abbiamo detto, consta di circa 1,3 miliardi. Sicuramente posso dire che sono stati meno interessanti i 300 milioni per le misure microsettoriali: non ci piacciono e non dovevano trovare spazio. Lo stesso ministro Tremonti le definì, a suo tempo, "un film dell'orrore" che non avrebbe voluto vedere più. Certamente dall'anno prossimo, con la

dei difensori civici), se estremamente positivo in termini di riduzione dei costi, sicuramente crea però problemi dal punto di vista dell'operatività degli enti locali e, soprattutto, determina una discrepanza che probabilmente ad un esame più attento in 1a Commissione, cioè nella sua sede naturale, avrebbe potuto trovare

non nascondiamocelo - sarebbe un segnale importante di solidità della maggioranza contro i *fan* della crisi permanente e delle elezioni anticipate.

della più grave recessione degli ultimi ottant'anni (perché di questo si è trattato). In estrema sintesi, il giudizio è che possiamo guardare con razionale fiducia al futuro del Paese.

hanno influito positivamente i giganteschi stimoli fiscali messi in atto da quasi tutti i Governi dei grandi Stati; ho detto «quasi» perché non tutti lo hanno fatto: uno di quelli che non li ha messi in atto è il Governo italiano. Terzo elemento che motiva quella razionale fiducia nel futuro: le famiglie dei Paesi emergenti potranno col tempo (ma non ci vorrà moltissimo, e questa è la novità positiva che emerge dai dati dell'economia globale) sostituire le famiglie americane come consumatori globali. In parte ciò è già avvenuto. C'è un dato impressionante nella situazione del 2009 in particolare: nelle vendite al dettaglio, le famiglie del BRIC - i quattro Paesi emergenti fondamentali - hanno già compensato la caduta delle vendite al dettaglio che si è determinata negli Stati Uniti d'America. È già così. Il quarto elemento che motiva quella fiducia nasce dal fatto che l'applicazione e la diffusione delle tecnologie pervasive

ha un sistema produttivo non spiazzato sotto il profilo merceologico dalle sue specializzazioni produttive. Pertanto, la diffusione e la produzione di queste nuove tecnologie possono aiutare il sistema produttivo italiano a mantenersi tra i grandi protagonisti dell'economia globale. A proposito dell'elemento rappresentato dalle potenzialità di consumo delle famiglie dei Paesi emergenti, vorrei citare qualche ulteriore dato perché nel dibattito pubblico italiano si tende a sottovalutare troppo questo elemento. Secondo gli andamenti attuali, nel 2030 il numero di coloro che nel mondo vivranno in condizioni di agio e di benessere è destinato ad aumentare di 420 milioni, aumentando di un terzo il numero delle persone agiate attualmente esistenti nell'economia globale. Per quell'anno - sempre il 2030 - 2 miliardi di persone in più si aggiungeranno a quelle che oggi compongono quella che chiamiamo classe media. c'è un elemento di fiducia nel futuro che emerge da questi dati, a mio avviso assolutamente straordinario. Abbiamo un sistema produttivo di beni, cioè siamo la manifattura d'Europa, e produciamo beni di qualità che piacciono alle persone che possono permetterseli, in tutto il mondo: entro il 2030 aumenteranno, fino ai livelli che ho richiamato. Vi è un ulteriore elemento che motiva la fiducia, da questo lato, nel futuro: sta aumentando, in particolare nei Paesi emergenti, il numero delle donne che partecipano alle forze di lavoro. Questo è un dato di modifica strutturale dell'economia globale, forse la più grande modificazione nell'economia globale di mercato che si sia conosciuta nel corso degli ultimi trent'anni. Questo vuol dire che ci sono redditi delle famiglie in aumento che si orienteranno verso consumi che sono quelli preferiti dalle donne. E noi abbiamo un sistema produttivo in grado di produrre beni che piacciono alle consumatrici globali, se hanno redditi tali da poterseli permettere. C'è un dato impressionante che viene dall'India, dove hanno dove hanno approvato recentemente una norma che in Italia chiameremmo «delle quote rosa»: hanno imposto per legge delle soglie per il numero di donne presenti nelle assemblee rappresentative.

sul terreno degli investimenti tali che - il dato è misurato da uno studio straordinario compiuto due economisti americani - addirittura abbiamo una situazione nella quale il governatore donna mediamente produce il 60 per cento di investimenti in più nel settore della potabilizzazione dell'acqua e del portare l'acqua potabile all'interno delle case rispetto ai governatori maschi. In sostanza, la presenza delle donne tra i decisori politici, poiché le donne cambiano la qualità dell'investimento e del consumo,

Naturalmente vi sono anche alcuni problemi. Il giudizio di fiducia razionale è fondato su elementi strutturali seri.

perché una brusca sterzata in termini restrittivi sia della politica di bilancio sia della politica monetaria potrebbe determinare il collasso della ripresa e il ritorno dell'economia mondiale in una situazione di recessione.

al livello di sviluppo del prodotto e della ricchezza nazionale precedente la crisi in quattro anni; gli Stati Uniti tornerebbero in un anno al livello di sviluppo del prodotto pre-crisi

negli Stati Uniti si tornerebbe a quel livello nel 2015 e nella Repubblica federale tedesca nel 2012. Questi dati, che sono estrapolati dall'attuale andamento dell'economia e della produzione industriale italiana e degli altri Paesi,

sarà costituita dal fatto che le decisioni di spesa delle famiglie e delle imprese troveranno per lungo tempo limiti seri nell'indisponibilità del credito necessario. Il contingentamento del credito è un dato strutturale

In Italia, come risulta dalla valutazione dei dati essenziali fornitici, per esempio, dal Fondo monetario internazionale, monetario internazionale, l'uso della politica di bilancio espansiva - c'è stato anche in Italia - è tutto da stabilizzatori automatici; gli strumenti fiscali discrezionali non sono stati usati in Italia. La manovra discrezionale è pari

adesso, nella fase della ripresa, al fatto che gli stabilizzatori automatici in automatico torneranno dove devono essere, perché le caratteristiche della spesa pubblica italiana e del nostro Stato sociale sono tali

sono - la forza di aggredire e sciogliere il nodo che stringe alla gola l'economia italiana e che risulta da questi due banali dati che vado a citare. Rispetto Rispetto alle previsioni, nel solo 2009 noi abbiamo risparmiato in spesa per interessi sul debito pubblico quasi 10 miliardi di euro,

sul versante del servizio del debito che, sapete bene, è una voce fondamentale della spesa pubblica italiana? Abbiamo aumentato di nuovo rispetto alle previsioni la spesa corrente primaria di quasi 7 miliardi di euro. È chiaro che così non si va da nessuna parte, perché così, naturalmente, abbiamo una politica che non riesce a suscitare nel Paese la necessaria fiducia nella possibilità di farcela, perché non fa bene il suo mestiere, perché non mette ordine in casa propria. La casa della politica, prima di tutto, è la pubblica amministrazione, è come si riesce a riqualificare, a rendere più efficiente e anche a ridurre il livello della spesa pubblica. Se non facciamo questa operazione e non innalziamo la produttività della spesa pubblica, non innalzeremo mai la produttività totale dei fattori e, quindi, non avremo una ripresa sostenibile nel tempo, duratura e significativa, potremmo avere se risolvessimo e affrontassimo questo problema. Da questo punto di vista, signor Presidente, la legge di bilancio e la legge finanziaria che discutiamo non sono dannose. Forse la manovra finanziaria danni non ne farà perché è certamente inutile: non affronta il nodo cruciale, così come potremo vedere esaminando gli emendamenti. Penso, per esempio, a quello del Gruppo del PD a proposito di impegno per ridurre la spesa corrente primaria, al fine di finanziare in automatico - e solo se si realizzano risparmi - con quei risparmi la riduzione dell'IRAP, riproponendo così una discussione che abbiamo fatto nel corso della prima lettura. Signor Presidente, abbiamo approvato sostanzialmente assieme, in quest'Aula, la legge sulla pubblica amministrazione, che non è la legge Brunetta - i membri del Governo lo sanno bene - ma la legge Brunetta-Ichino. Allora, qual è la proposta che noi avanziamo? Questa è la prima proposta che avanziamo: abbiamo una legge sostanzialmente approvata assieme; associamo all'attuazione di quella legge risparmi di spesa puntuali e crescenti nel tempo e, in quanto si realizzano quei risparmi finanziamo interventi di riduzione mirata e selettiva della pressione Questa è la prima base di un intervento che cambierebbe profondamente la politica di bilancio di questo Paese e renderebbe il sistema Paese più produttivo, agendo dal lato che in questo momento penalizza il sistema Italia, che non è vero che non ha imprese capaci di competere nel mondo e lavoratori ingegnosi e impegnati a sufficienza. Ha tutto ciò, ma ha anche una politica che non fa il suo mestiere e non è capace di fare la propria parte (purtroppo si può dire, in una certa misura, persino indipendentemente dalle maggioranze che *pro tempore* governano). A questo abbiamo fatto seguire nel corso della discussione in Commissione puntuali e precise proposte d'intervento, selezionando quelle che magari oggi, dal punto di vista quantitativo, possono non avere le dimensioni necessarie per imprimere una svolta, essendo qualitativamente strategiche, rendono la politica in grado di interloquire con il Paese producendo fiducia, invece che alimentando la sfiducia come sta accadendo

è quello con la minore partecipazione delle donne alle forze di lavoro, aspetto che si concentra in particolare nelle aree dell'Obiettivo 1. Cosa proponiamo? Cosa sarebbe necessario? Ridurre la pressione fiscale sul lavoro femminile, Ridurre la pressione fiscale sul lavoro femminile, in maniera da rendere più conveniente per un'impresa assumere una donna a parità di lavoro, di prestazione, di salario e di produttività rispetto ad un lavoratore maschio. Solo così si riequilibrano le opportunità a favore delle donne e si utilizza la principale risorsa oggi inutilizzata dal Paese per il suo sviluppo, rappresentata dalla qualità e e dalla quantità di giovani donne in età di lavoro che non vanno sul mercato del lavoro perché sono sfiduciate circa la possibilità di trovarne uno legale. Si può cominciare piano, concentrandosi molto sulle aree dell'Obiettivo 1 o solo su alcune aree dell'Obiettivo 1,

- che riguarda la mobilità del fattore lavoro. La crisi - diceva un maestro come Schumpeter - è la sede per la distruzione creatrice: vi sono imprese e posti di lavoro che non reggono;

se ragioniamo su questo punto, vediamo come la distruzione creatrice si può realizzare se c'è la mobilità del fattore lavoro; ma se il trattamento fiscale degli affitti oggi è tale da rendere impossibile che il mercato degli affitti il mercato degli affitti sia agibile, il proprietario della casa, che dovrebbe cambiare posto di lavoro e andare in un'altra parte del Paese, non riesce ad affittare casa sua, quindi non riesce ad affittarne un'altra per sé là dove ci sarebbe un lavoro che potrebbe fare. Risultato? Sta fermo dov'è, a causa del non funzionamento del mercato degli affitti. Cedolare secca, detrazione su chi paga l'affitto, cedolare secca sull'affitto percepito: ecco la soluzione che farebbe emergere il nero - e questo è certamente vero, com'è assodato da tutti - ma che soprattutto favorirebbe la mobilità del fattore lavoro sul territorio.

a fare la nostra parte di grande partito che vuole sostituire il PdL, che appare senza coraggio e senza determinazione nel perseguire una strategia di riforme. Ed è per questo che, anche dall'opposizione, pensiamo di dover fare e di riuscire a fare pienamente la nostra parte. *(Applausi dal Signor Presidente, rappresentanti del Governo,

che il peggio sia passato ma che vi sia ancora una crisi molto lunga da superare, una crisi pesante, che genera una grande preoccupazione, in particolare fra molti strati sociali del nostro Paese. L'interrogativo che quasi tutti o comunque gran parte dei cittadini che abbiamo incontrato ci ha posto è cosa succederà dopo questa crisi, cosa sarà del nostro Paese, o meglio, come usciamo da questa crisi,

Per la prima volta abbiamo avuto netta la sensazione che stia succedendo qualcosa di profondo nel cuore della gente che abbiamo incontrato peraltro, non ci dice mica che la ricetta giusta è quella nostra; non ci dice ancora questo. Ci dice, però, che le ricette del Governo non vanno bene, che non sono sufficienti, che sono inadeguate.

la gente, il nostro Paese ci interroga in questo modo. D'altra parte, se la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia comincia a sostenere che serve un progetto per il futuro del nostro Paese e se il governatore della Banca d'Italia Draghi afferma che servono riforme, a partire da quella degli ammortizzatori sociali, una ragione ci sarà e noi crediamo che ci sia. Qual è, allora, la nostra proposta alternativa? Sì, alternativa a quella del Governo. Noi ne indichiamo una davvero

prima di tutto il Patto di stabilità con quattro, cinque miliardi da mettere a disposizione degli enti locali. Cosa vi costa fare un'operazione seria e chiara? Quelle che finora sono state fatte non sono chiare, non funzionano e non danno impatto.

Ci sono 10, 12, 15, 17 miliardi (qualcuno dice che siano molti di più) che non girano, e non girano nelle imprese del nostro Paese. In tal modo la pubblica amministrazione non paga, le imprese non pagano i fornitori e accade che oggi tutti si lamentano. C'è una situazione che sta mettendo a repentaglio le imprese più esposte e che, anche se hanno lavori e commesse, sono in grande difficoltà. La terza questione su cui

per cento; rimettetela sul risparmio energetico: farete cosa buona e utile per aprire dei cantieri. E di questo oggi abbiamo bisogno.

dopo il federalismo fiscale non ci si può fermare. Da lì bisogna andare avanti: è veramente in ballo la nostra credibilità, ma anche la vostra!

proposte, ad esempio sulla riforma della contabilità; siamo pronti a misurarci con voi per dare un segnale - in questo caso, sì - vero di fiducia al Paese. Ho citato gli elementi più significativi ma l'idea che ci siamo fatti è quella di un Paese che ci chiede: cosa fate lì se non fate nulla per riformare un Paese vecchio, che ci tira indietro? Questo ci dicono tutti gli imprenditori: ci tira indietro e non ci spinge verso il futuro.

anche ragione. Superare il bicameralismo, riformare il sistema istituzionale, i sistemi di rappresentanza, le prefetture, le camere di commercio: se giriamo attorno alla spesa pubblica, per togliere un po' di burocrazia ed affrontare davvero l'organizzazione dello Stato in questo Paese, delle risorse ce ne sono, e tante. Bisogna avere la volontà

sostegno alle famiglie ed ai redditi, cedolare secca sugli affitti. Sono proposte responsabili, che trovano una larghissima condivisione anche nella vostra maggioranza.

che investono in ricerca e innovazione, a quelle che creano posti di lavoro e che aiutano i giovani e le donne, in particolare, ad inserirsi nel mondo del lavoro. Come diceva il senatore Morando, le risorse andrebbero

Con i nostri emendamenti abbiamo quindi messo in campo una proposta alternativa per il Paese, alternativa alle pezze,

una proposta alternativa alla vostra, più in sintonia con il Paese e, secondo noi, anche più efficace. Se davvero, infine, volete dialogare e confrontarvi,

serie, che sicuramente possono aiutare questo Paese, e rispetto alle quali noi continueremo ad incalzarvi e a tenere alta l'iniziativa. Signor Presidente, colleghi, il Senato è chiamato a trattare in terza lettura la finanziaria approvata dalla Camera

delle misure che la Commissione bilancio della Camera ha consegnato all'Assemblea, come le ha puntualmente ricordate il nostro relatore senatore Saia. Si tratta di misure che afferiscono a settori specifici, a nostro a nostro avviso importantissimi, come il *welfare*, lo sviluppo economico, le infrastrutture, la pubblica amministrazione e gli enti locali. Sono misure che hanno portato ad una modifica significativa dell'ammontare complessivo di questa manovra: per il prossimo anno è di circa 9 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e di oltre 5 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, a fronte delle limitate modifiche alle cifre originarie determinate in prima lettura da questo ramo del Parlamento, segno del grande controllo di questa finanziaria sulla tenuta della finanza pubblica. Ma queste diversità non devono considerarsi conseguenti ad uno stravolgimento dell'impostazione che ha caratterizzato originariamente la manovra finanziaria. Mi sono sembrate immotivate, in tal senso, le polemiche che hanno accompagnato i lavori nell'altro ramo del Parlamento, che tendevano a descrivere quei lavori come un *blitz* (io non credo sia possibile affermare

questa maggioranza sostiene essere, ormai e fortunatamente, un lontano ricordo. Vorrei ricordare che già in corso di prima lettura il ministro Tremonti in quest'Aula aveva chiaramente preannunciato significative modifiche successive, possibili in ragione dell'ammontare, che si sarebbe determinato con il passare dei giorni, delle entrate prevedibili a seguito della regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero grazie allo scudo fiscale. E mi sia consentita una piccola digressione al riguardo: lo scudo si è rivelato un provvedimento importante, che ha mantenuto le promesse logiche e strutturali sulle quali era stato congegnato, quello di assicurare risorse all'economia. Un successo per il quale, non a caso, ne è stata decisa la proroga. Come dicevo, le innovazioni introdotte dalla Camera non sono state quindi il frutto di un *blitz* insensato, la decisione di creare tanti, quanto inutili, rivoli di spesa. Le innovazioni, al contrario, rientrano nella stessa logica che ha animato l'originaria impostazione di questa manovra: la prudenza, quella prudenza fiscale che in una situazione di crisi ed incertezza dell'economia globale - il cui punto più alto sembra superato, ma che non è ancora possibile dire che è definitivamente alle nostre spalle - è stata responsabilmente perseguita dal Governo. Sin dal luglio 2008, l'Esecutivo ha sempre dichiarato di voler contrastare gli effetti negativi della crisi, adottando misure specifiche a sostegno di vari settori o situazioni sociali, tutte sotto il vincolo dell'impatto il più possibile neutrale sulla finanza pubblica. Superfluo, ormai, ripetere la preoccupazione per i rischi connessi ad un peggioramento del disavanzo per un Paese su cui grava un debito pubblico, in rapporto con il prodotto nazionale, delle dimensioni che tutti, purtroppo, conosciamo. E la promessa è stata ancora mantenuta. Come non dire che le misure approvate dalla Camera sono "a sostegno"? Penso a quelle che prorogano gli ammortizzatori sociali e li estendono ad altri beneficiari (i lavoratori a progetto), a quelle per le imprese (come i crediti di imposta per l'innovazione o la partecipazione della Cassa depositi e prestiti a fondi di finanziamento e sviluppo per le piccole e medie imprese), a quelle relative alla Banca del Mezzogiorno (finalizzate ad una sinergia tra banche e sistemi finanziari ed all'incremento delle infrastrutture), a quelle sui Confidi. Sono tutte misure a sostegno di aspetti sociali e dello sviluppo economico, in un *mix* con altri interventi: dalla sperimentazione della cedolare secca sugli affitti (ciò in vista anche del federalismo fiscale), ai buoni libri, alla sicurezza scolastica, alla gestione e responsabilizzazione dei deficit sanitari, alle misure che riguardano il funzionamento dello Stato e degli enti locali. Una serie di misure che hanno portato ad una significativa ricomposizione del quadro contabile delle entrate e delle spese, ma che - come è stato messo in evidenza anche dalla documentazione prodotta dagli Uffici della Camera - hanno lasciato sostanzialmente invariati gli effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al testo approvato dal Senato. Un'impostazione, questa, testimoniata dai quadri della legge dì bilancio e dagli allegati di quella finanziaria. Da dove, peraltro, emerge chiaramente un aspetto che mi sembra vada giustamente evidenziato: quella che si sta per chiudere è una manovra improntata alla qualità degli interventi qualità, prima ancora che alla quantità), realizzati senza aumentare la pressione fiscale e le tasse. Una particolarità non proprio irrilevante e non proprio facile da perseguire che consente di pensare con minore pessimismo - speriamo Io voglio ricordare, a me stessa e a tutti noi, che la nostra presidenza del G8 tenutosi all'Aquila qualche mese fa, aveva un preciso titolo: «La persona prima di tutto»; "*People first*", dicemmo ai Paesi che si interrogavano con noi su come uscire da questa drammatica crisi. Ebbene, questa è la finanziaria dedicata a quelle persone, a quei cittadini italiani e a quelle cittadine italiane che usciranno da questa crisi grazie agli interventi di protezione, e di sviluppo al contempo, che questo Governo è riuscito e riuscirà a garantire anche con questa finanziaria. *(Applausi

abbiamo espresso un giudizio molto negativo su questa finanziaria *light*, perché essa non risolve nessuno dei problemi del Paese: né quello del debito pubblico (che ha sfondato il muro dei 1.800 miliardi di euro), né quello della disoccupazione (che continua a crescere), né le altre grandi questioni. Qualche giorno fa, c'è stata una stima sui pignoramenti e sulle esecuzioni immobiliari che aumentano, nell'ultimo triennio, del 60,5 per cento. Non si dà alcuna risposta

sono peggiorati fra il 2008 e il 2009 di circa 44 miliardi, attribuibili solo per 10 miliardi a un calo delle entrate (soprattutto di quelle tributarie). I restanti 34 miliardi sono tutti legati a un incremento della spesa primaria, che aumenta del 5 per cento in termini nominali (2,7 in termini reali). Se poi guardiamo alla composizione degli incrementi della spesa, ci rendiamo conto che sono quasi tutti concentrati nella spesa pensionistica

in parte (quasi 2 miliardi) per il riacquisto, imposto all'lNPS, di immobili cartolarizzati con le operazioni SCIP1 e SCIP2 (varate sempre dal ministro Tremonti) per evitare il fallimento della società cui erano state affidate tali iniziative. I nodi vengono sempre al pettine. Anche nel 2010, secondo i conti previsionali dell'INPS, i contributi previdenziali dovrebbero diminuire. Insomma, questa finanziaria non risponde ad alcuna delle questioni del Paese. Ci sono alcuni contributi dati dati per finanziare le clientele; mi riferisco ai 130 milioni per gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, ai 370 milioni di euro per la stabilizzazione,

proroga per le agevolazioni fiscali, eccetera. C'è una crisi profonda che attraversa il tessuto sociale che bisognerebbe affrontare. L'ultimo rapporto CNEL sul sovraindebitamento delle famiglie a rischio usura ritrae una realtà divisa in quattro quarti: un quarto di famiglie ha migliorato il proprio reddito, un quarto, seppur con qualche difficoltà, riesce a cavarsela, due quarti invece vedono peggiorare la loro condizione con una situazione preoccupante specie per gli anziani. In tale contesto cresce solo la raccolta di giochi e scommesse che, nel 2010, potrebbe raggiungere i 58 miliardi, pari al 3,7 per La raccolta complessiva nei primi nove mesi del 2009 ha superato infatti i 39 miliardi (+14,4 rispetto ai primi nove mesi del 2008), con valore medio di raccolta mensile di 4,3 miliardi di euro e punte massime di 4,5 miliardi di euro registrati nei mesi di gennaio e marzo. Il *trend* di crescita potrebbe quindi proseguire per raggiungere quella somma. È da molto tempo che chiediamo al Governo di agire per affrontare i gravi disagi sociali e per ridurre l'enorme massa del debito pubblico seguendo politiche di tagli a sperperi, sprechi e finanziamenti a fondo perduto (che nel 2009 si attestano a ben 39 miliardi di euro), mediante la vendita di oro e riserve della Banca d'Italia (pari a oltre 72 miliardi di euro ai valori correnti), coerentemente alle dismissioni delle riserve auree effettuate da tutti i Paesi dell'Eurozona, nonché alienando il patrimonio demaniale e gli immobili non più necessari alle pubbliche amministrazioni. Il Governo, tuttavia, ha preferito impegnare molti miliardi per ridurre l'ICI a chi non ne aveva bisogno e per addossare il salvataggio dell'Alitalia a carico della fiscalità generale, piuttosto che adottare azioni concrete di contenimento del debito, che, nonostante i tassi in discesa, si dovrebbe ridurre meccanicamente per i minori interessi. Ora i nodi vengono al pettine e su 8,9 miliardi di euro, ben 2 devono essere destinati a SCIP1 e 2, per evitarne il fallimento. Invece di contrastare l'evasione si approva lo scudo fiscale, una premialità di vantaggio per i disonesti che continueranno a vivere sulle spalle degli onesti, per sbiancare ciclicamente i capitali per la terza volta dal 2001 nella grande lavanderia statale, per evadere e frodare il fisco, certi di farla sempre franca. Per queste ragioni, noi dell'Italia dei Valori non possiamo condividere un impianto di finanza pubblica che non affronta i problemi del Paese, che va a scippare ben 3,1 miliardi di euro del TFR, del TFR, che sono soldi dei lavoratori, e non affronta i problemi della ricerca (come è stato appena ricordato, ci sono quattro lavoratori che sono saliti per denunciare la minaccia di licenziamento); non affronta neppure la cassa integrazione, né la distruzione della ricchezza ad opera di banchieri con i quali il Governo continua ad andare a braccetto, certi di non pagare mai il conto per i disastri provocati e che possono continuare a brindare con *champagne* di marca con i *bonus* percepiti sulla pelle di pensionati al minimo, di lavoratori, casalinghe e piccole e medie imprese artigiane strozzate e massacrate dalla stretta creditizia e dalla distruzione del sudato risparmio.

delle famiglie e dei contribuenti. Deve essere allora un refuso, signor Presidente, il comma 200 che autorizza, a decorrere dal 2010, anticipazioni tariffarie di tre euro a passeggero in favore di quei capitani coraggiosi, di quei gestori aeroportuali, configurando una vera e propria stangata tariffaria a carico dei viaggiatori, tanto per far uscire il settore dei trasporti dalla gravissima crisi. Deve essere un ulteriore errore il comma 215 sulle spese di giustizia, in particolare il contributo unificato pari a 103,3 euro a carico dei lavoratori licenziati che fanno ricorso in Cassazione. Sarà certamente un altro sbaglio il comma 6-*bis* dello stesso articolo, che introduce un ulteriore balzello, pari ad un contributo minimo di 38 euro a carico di quei cittadini

signori della maggioranza, non potremo votare una finanziaria che occulta sapientemente tasse e balzelli e che non risolve alcuno dei problemi del Paese, neanche con misure temporanee,

quella che andiamo ad esaminare è una finanziaria a dir poco di basso profilo: giornalisticamente è stata definita una finanziaria di "galleggiamento", e per di più è, paradossalmente, costosa. È stato detto più volte che la finanziaria sarebbe stata un ottimo veicolo per introdurre importanti riforme. La prima riforma, quella che andava fatta fin dall'inizio della recessione, avrebbe dovuto essere quella degli ammortizzatori sociali, che avrebbe permesso all'Italia di uscire in maniera molto più efficace da questa situazione di recessione. Avrebbe dovuto quantomeno essere una finanziaria utile a far riemergere l'economia nazionale, se non dall'attuale situazione, almeno da quella stagnazione in cui la nostra economia si è trovata prima dell'esplodere della crisi. In una situazione così seria si sarebbero dovuti predisporre dei programmi, dei progetti per rilanciare l'economia. Inizialmente il Governo aveva parlato di grandi piani, a partire da quello per la rinascita del Sud, ma di questi grandi piani si è persa ogni traccia e sono totalmente assenti in questa finanziaria. Le risorse del provvedimento sono ricavate sostanzialmente da due grandi voci. La prima è lo scudo fiscale, che dovrebbe favorire il rientro in Italia dei capitali illegalmente esportati all'estero; la seconda è il versamento da parte dell'INPS, nel bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (TFR). Certamente si tratta di operazioni legittime da un punto di vista giuridico, ma entrambe altamente censurabili sul piano politico e su quello degli effetti economici pratici. Lo scudo fiscale non può che essere definito ancora una volta un atto di pura e semplice inciviltà: infatti premia, non solo chi ha evaso le tasse, ma chi spesso ha commesso anche altri reati. dunque, oltre ad essere un condono, secondo noi dell'Italia dei Valori, è un'amnistia. Per quanto riguarda lo spostamento in bilancio del TFR, si tratta di un modo per ritornare a pratiche di contabilità creativa di cui non si sentiva proprio la mancanza e che dovevano essere assolutamente abbandonate, sia perché hanno già dato pessimi risultati in passato, sia perché sono totalmente inadatte in una fase di crisi così pesante. di un'operazione pericolosissima, che crea debito pubblico, accentua il disavanzo e, peraltro, è passibile di censura da parte dell'Europa. Conosciamo l'obiezione sollevata da più parti: l'utilizzo delle risorse del TFR era già stato posto in essere dal Governo Prodi. Peccato, però, che chi solleva tali argomenti lo faccia in maniera incompleta, facendo finta di dimenticare che la famosa norma contenuta nella finanziaria per il 2008 prevedeva un intervento limitato nel tempo, e che le risorse in questione venivano destinate esplicitamente a specifici investimenti. Di fatto, invece, quanto previsto all'articolo 2, 2, comma 105, del provvedimento attuale si risolve in un prestito forzoso che i lavoratori fanno allo Stato per coprire la spesa corrente, peraltro senza che sia posto alcun obbligo in capo al Governo di rendere conto circa l'utilizzo effettivo delle risorse o i tempi di restituzione delle stesse. Per quanto concerne il lavoro, come sottolineato all'inizio, il Governo oltre a non porre in essere alcuna riforma vera, non adotta neppure quei provvedimenti semplici, ordinari, poco costosi che potrebbero offrire riparo dagli effetti della crisi ad un maggior numero di persone. Anzitutto la proroga della cassa integrazione ordinaria per le grandi imprese, visto che le risorse ci sono: un tale provvedimento permetterebbe, attraverso l'utilizzo dei fondi della cassa integrazione più volte sbandierati dal Governo in carica, di dare una minima certezza ai lavoratori per il futuro. Sarebbe necessario, inoltre, considerare il fatto che c'è una parte di lavoratori che non beneficiano della cassa integrazione (neppure di quella in deroga), e per i quali la situazione si fa sempre più difficile. Infatti, anche chi ha percepito l'indennità di disoccupazione ormai la sta esaurendo e, in base alla normativa attualmente in vigore, si vedrà purtroppo impossibilitato a richiederla nuovamente perché, non avendo lavorato nell'anno precedente, non ne ha più i requisiti. Le risposte della finanziaria ai suddetti problemi o non ci sono o vanno nella direzione opposta. Si scarica semplicemente sulla cassa integrazione in deroga anche il peso delle grandi imprese che finiscono la cassa integrazione ordinaria. invece prevista la reintroduzione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto *staff leasing*), che si è dimostrato, nella pratica, il principale generatore di precarietà del nostro mondo del lavoro. La sua reintroduzione non era stata richiesta da nessuno ed era stato peraltro abolito nel 2007 dal Protocollo sul *welfare* con il consenso di tutti; dunque, non si capisce il motivo della sua reintroduzione, se non per il semplice fatto di voler penalizzare ancora un volta i lavoratori. Insomma, una pura provocazione politica. Allo stesso modo si deve leggere la norma contenuta nel comma 212 dell'articolo 2, che elimina l'esenzione dalla corresponsione, a carico dei lavoratori, del contributo unificato nelle cause di lavoro, previdenziali ed assistenziali, dinanzi alla Corte di cassazione. Si tratta di una norma assolutamente irrazionale, dato che è prevista l'esenzione nei primi due gradi di giudizio, e che avrà il risultato di ridurre, di fatto, la possibilità del ricorso di ogni lavoratore dinanzi alla Cassazione. Quantomeno incomprensibile è anche la scelta di destinare le risorse per la ricollocazione dei lavoratori alle agenzie interinali, anziché alle imprese che assumono; una scelta davvero strana, visto che uno dei pochi incentivi che ha sempre funzionato è stato quello volto a premiare chi assume dalla mobilità o dalla disoccupazione, creando posti di lavoro a tempo indeterminato. Ancora, si sceglie la via, puramente di facciata, della proroga dei contratti di produttività in un momento di crisi produttiva, e non si interviene invece, ad esempio, con una detassazione delle tredicesime, che, aumentando il potere d'acquisto delle famiglie, faccia davvero ripartire i consumi e, di conseguenza, l'economia. Infine, si taglia di ben 100 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 2, comma 158): ancora una volta tagli laddove ci sarebbe bisogno di investimenti. Il Governo, purtroppo continua a Governo, purtroppo continua a comportarsi come se l'Italia non avesse subito la crisi e non avesse bisogno di far ripartire l'economia. Pertanto, il nostro voto non può che essere nettamente contrario.

un nuovo atteggiamento da parte della maggioranza, sia alla Camera che al Senato. Invece, questo non c'è stato. Si deve discutere anche di questo episodio,

interventi di ordine addirittura personale presenti in questa finanziaria, oltre al rilancio della legge mancia. Viva la Lega, che spesso ci ha fatto da da moralizzatrice in quest'Assemblea! Ritorna la legge mancia e addirittura mi consta che alla Camera la Commissione ha già deliberato quali devono essere i criteri di divisione.

di quella politica promessa che doveva rilanciare il Mezzogiorno come questione di ordine nazionale, abbandonando quelle politiche di clientele che tutti respingiamo.

va benissimo dopo 40 anni, ma è necessario dare una risposta di ordine globale che fissi il diritto dei popoli e delle comunità. La ricostruzione non può essere legata

Non è possibile - l'ho detto tante volte - strumentalizzare la sofferenza, esporre la sofferenza ai vari *gossip*. Alle calamità si risponde con la solidarietà generale di un popolo. La solidarietà generale di un popolo dice che bisogna trattare tutti alla stessa maniera: dal Nord al Sud.

I dati di ottobre 2009 evidenziano una leggera ripresa del PIL. Nonostante la forte diminuzione delle entrate fiscali dei primi mesi, gli ultimi dati sul gettito tributario rilevano che l'Italia è il Paese, in Europa, che ha tenuto meglio e con la minore contrazione delle entrate tributarie (meno 3,4 per cento nel periodo che va da gennaio a ottobre). Quasi tutti gli altri Paesi presentano tassi di variazione negativi superiori al 10 Questi, cari colleghi dell'opposizione, sono dati non parole. Il nostro Paese ha tenuto meglio di molti altri, questo dato è incontestabile. Ciò è avvenuto grazie all'efficace azione del Governo, Governo, al minore debito privato e al lavoro delle nostre piccole e medie imprese che fanno della flessibilità e della continua innovazione la loro grande forza. forza. Stiamo per mandare in archivio un 2009 che per il nostro movimento è stato certamente positivo. I tanti importanti risultati ottenuti grazie alla quotidiana azione dei nostri Ministri, dei nostri parlamentari a Roma e dei nostri amministratori locali sul territorio sono sotto gli occhi di tutti. Basti pensare al drastico calo (meno 90 per cento) degli sbarchi di clandestini, all'aumento della sicurezza nelle nostre città, al federalismo fiscale che il Parlamento ha approvato definitivamente e alla difesa e salvaguardia delle nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medie, dei nostri posti di lavoro e della nostra economia in un periodo di pesante crisi finanziaria internazionale che ha colpito tutti i Paesi occidentali. ancora alla protezione e alla valorizzazione del lavoro dei nostri allevatori e agricoltori, alla battaglia che ha permesso di introdurre il marchio DOC *made in Italy* per tutelare i nostri prodotti oppure, per quanto concerne la lotta agli sprechi, il taglio di quasi 40.000 leggi inutili e l'approvazione del codice per le autonomie. Una politica invece che si basasse su di un considerevole aumento della spesa pubblica, come richiesto a gran voce dall'opposizione, porterebbe ad annullare gli effetti positivi delle manovre anticrisi e ad un progressivo aumento degli interessi passivi sul debito

Nel 2010 questi interventi interesseranno 45.000 aziende e 250.000 lavoratori per il mantenimento della forza lavoro e per il sostegno delle nostre aziende. Sempre in campo di *welfare* siamo intervenuti con la definizione del patto sulla salute, che sarà la vera sfida per le Regioni e che apre la strada alla grande sfida che si chiama costo standard e federalismo. Per le Regioni che sforano, che creano i buchi nella sanità, si prevede una maggiorazione delle tasse regionali che ricadranno sui loro cittadini e che potranno pertanto, con il loro voto, mandare a casa per sempre i politici che creano per incapacità e malafede i dissesti sanitari. poi 24 miliardi per l'edilizia sanitaria, in un Paese che ne ha sicuramente bisogno, e 400 milioni per i fondi per la non autosufficienza. E che dire degli interventi per la scuola? La legge finanziaria prevede un fondo di 300 milioni per la messa in sicurezza dei plessi scolastici, che saranno immediatamente disponibili e cantierabili. Abbiamo inserito, sempre in tema di scuola, un finanziamento di 103 milioni per il contributo alla gratuità dei libri, di 130 milioni per il finanziamento della scuola paritaria (molte delle scuole paritarie sono cattoliche e svolgono un importante ruolo educativo dei nostri ragazzi, in quanto sono il baluardo dell'autonomia scolastica) e di 400 milioni per l'università. Abbiamo rifinanziato nella misura di 400 milioni il 5 per mille per le associazioni di volontariato.

a muovere da una forte ricapitalizzazione dello strumento del credito d'imposta per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo: più di un miliardo è stato messo a disposizione del sistema delle imprese.

Agli enti locali - è vero - non siamo riusciti a dare tutte le risposte, ma non possiamo negare di aver trovato le risorse per rimborsare l'ICI ai Comuni (156 milioni per il 2008 e 760 per il 2009): è stato un importante riconoscimento da parte del Governo del ruolo fondamentale per l'erogazione dei servizi essenziali che svolgono gli oltre 8.000 Comuni d'Italia, anche se - come saprà, signor Vice Ministro - rimane irrisolto il tema del Patto di stabilità degli enti locali,

Per la sicurezza, sono stati stanziati 500 milioni per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri: altro che indulto, noi scegliamo la strada di costruire nuove carceri! Per la Polizia e i Vigili del fuoco abbiamo previsto fondi per assunzioni a tempo indeterminato per 115 milioni nel 2010, per 344 milioni nel 2011 e per altri 600 milioni a decorrere dal 2012. Abbiamo garantito il *turnover* per le forze di polizia e per i Vigili del fuoco: alla faccia dei tagli alle forze di polizia e alla sicurezza che dichiara la sinistra!

Per questi e altri qualificanti motivi, che avremo modo di riprendere in altri momenti, possiamo dire di essere soddisfatti e di aver lavorato bene anche in questa finanziaria,

E nel 2010 che sta per iniziare, oltre a proseguire in questo cammino di cambiamento e di riforme, continueremo a combattere, con l'energia e l'ostinazione che da sempre contraddistinguono noi della Lega Nord e il nostro segretario Umberto Bossi, le nostre battaglie storiche in difesa della nostra identità, delle nostre tradizioni, della nostra economia e delle nostre famiglie. Vorrei infine ringraziare il presidente Azzollini, i relatori, il vice ministro Vegas, i componenti di maggioranza e opposizione, i tecnici ed i funzionari per il pregevole lavoro che abbiamo svolto in Commissione. PRESIDENTE.

generale. Abbiamo scelto di concentrare il poco tempo a disposizione per illustrare le nostre concrete proposte di correzione della manovra. Non posso, tuttavia, fare a meno di sottolineare una forte anomalia nella procedura che è stata seguita anche per l'approvazione di questa legge finanziaria. Basta citare il seguente dato: il testo che è uscito dal Senato prevedeva degli oneri di copertura pari a 765 milioni di euro; il testo che ci viene restituito dalla Camera porta oneri per 17,3 miliardi di euro. Quindi, non c'è nessuna parentela tra i due

si finisce per annegare ogni volontà, ogni direttrice di marcia. Di nuovo è la fiera degli interventi localistici, microsettoriali, ordinamentali

che questo provvedimento avrà nel far fronte alla crisi del nostro Paese. I dati italiani li conosciamo; li conoscete, colleghi. Mi permetto solo di ricordare quelli che riguardano la mia regione, il Veneto,

calo del prodotto regionale di oltre quattro punti e mezzo. È il risultato peggiore dal dopoguerra: non c'è mai stato un anno, dalla fine della seconda guerra mondiale, in cui ci sia stato un calo di queste dimensioni del prodotto regionale.

con l'azione di politica economica ad aiutare l'aggancio di questa ripresa e ad accelerare, perché non è scontato che questo avvenga com'è avvenuto per il passato;

sulla sua qualità soprattutto sotto due profili. Il primo è quello della capacità di individuare con nettezza le priorità necessarie: se le risorse sono poche, alla politica spetta scegliere con nettezza.

riguarda il lavoro, non posso negare che in questa finanziaria c'è la scelta da parte del Governo di destinare risorse cospicue, rispetto alle possibilità, in direzione di un cosiddetto pacchetto lavoro. Si tratta un miliardo e 100 milioni di euro; si tratta di notevoli risorse, però, se lo esaminiamo dal punto di vista delle priorità, ci accorgiamo che i nove decimi di questo pacchetto sono destinati ad incentivare la contrattazione di secondo livello, finalità che condividiamo perfettamente; così come l'abbiamo proposta, abbiamo condiviso la scelta del Governo e pensiamo che sia uno strumento importante di ammodernamento del mercato del lavoro. Ma non può succedere che

*una tantum* di qualche centinaio di euro; l'utilizzo dei fondi del trattamento di fine rapporto ricordo che la scelta del Governo Prodi, aspramente criticata dall'allora minoranza ora maggioranza, ha garantito circa

interventi ripetitivi nel tempo con fondi che sono dei lavoratori ed andrebbero mantenuti nel circuito della produzione di ricchezza economica. l'indicazione di priorità delle azioni contro la povertà; non voglio sostenere che l'Italia è diventata tutta povera. Il problema dell'Italia è la forte disparità sono certamente dei ceti, dei gruppi sociali che non hanno avvertito in modo drammatico il mordere della crisi; ma c'è una parte del Paese che sta soffrendo e per questa parte non vi è nessun un intervento. Ricordo che la famosa «Carta degli acquisti», che avrebbe dovuto raggiungere 1,3 milioni di cittadini italiani, attualmente viaggia su un utilizzo di circa 450.000 persone perché le caratteristiche di esclusione previste dal Governo impediscono di avere un intervento efficace sulle nuove povertà. Il secondo aspetto è il tema del clima. Ebbene, il Governo è reduce da impegni molteplici, assunti nei massimi organismi internazionali: prima il G8 a L'Aquila, poi il G20 a Pittsburgh; infine, la Conferenza sul clima a Copenaghen. La domanda è: che rispondenza c'è tra questi impegni assunti e la realtà delle azioni previste dalla legge finanziaria? in quanto nessuno di quegli impegni solenni si è tradotto in una posta della legge finanziaria, in un'azione innovativa. Anzi,

oggi ad alta profittabilità. Vi è una base produttiva italiana che sta reggendo la concorrenza internazionale; ci sarebbero tutti i motivi per sostenere investimenti in questa direzione, invece, si toglie quel che c'è. Capisco la difficoltà di raggiungere gli obiettivi di Kyoto in un momento difficile per il sistema industriale, ma allora concentriamoci sulle altre voci che intervengono positivamente sulla riduzione dei gas serra, serra, su efficienza e risparmio energetico, sulle tre grandi voci (trasporti, rendimento energetico degli edifici, fonti rinnovabili). Invece, cosa fanno la legge finanziaria ed il bilancio? Sui trasporti ricordo che la missione «diritto alla mobilità» vede diminuire gli stanziamenti del 18 per cento; gli investimenti per la mobilità locale calano del 25 per cento; gli investimenti sul sistema ferroviario passano da 5,5 miliardi a circa 3 miliardi di euro e poi ci meravigliamo di quello che succede nel Paese di fronte ad una nevicata? Avete eliminato l'intervento di agevolazione del 55 per cento sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici, edifici, a danno di tutta una filiera di piccolo lavoro artigiano che ha avuto un ruolo molto importante nel sostegno dell'economia in questo settore. le bioenergie, ricordo che avete eliminato lo stanziamento di 160 milioni di euro a favore delle produzioni

Approfitto per ricordare, a questo proposito, che una parte degli interventi previsti a Copenaghen passano per interventi di cooperazione internazionale a favore dei Paesi meno

il ministro Tremonti, che è molto efficace nella sua comunicazione, non abbia trovato altra chiave di lettura per presentare la legge finanziaria che quella di esaltare lo scudo fiscale: ci ha detto il Ministro che si tratta di una colossale manovra di potenziamento della nostra economia, perché i capitali che erano fuori tornano in Italia e servono per tenere aperte le imprese, non licenziare e gestire i rapporti tra creditori e debitori. Ma è proprio vero questo? Io penso di no. Innanzi tutto si tratta, in senso tecnico, di un vero e proprio condono. Questo provvedimento ha tutte le caratteristiche del condono perché permette di non pagare le imposte evase. evase. Al condono si accompagna una vera e propria amnistia di gravi reati penali. Ricordo che i condoni sono una delle tante forme di indebitamento di uno Stato: si incassano dei soldi subito perdendo la possibilità di incassarne di più in futuro. Come sempre, il condono porta con sé l'aspettativa di un altro condono, e difatti si è prorogato il termine. Come ci ha ricordato il gruppo degli economisti il ministro Tremonti ha rilasciato questa dichiarazione: «Chi continuerà a tenere i soldi in Svizzera, sappia che sono soldi morti».

ed è difficile che questi soldi vengano investiti. C'è poi una parte che riguarda la pulitura di capitali malavitosi;

ma l'aumento del controllo criminale sull'economia italiana. Infine, ci sono soldi reali che stavano nei paradisi fiscali; ma capitali che in tre mesi rientrano in Italia difficilmente appartengono

e la regolarizzazione ad un impegno di investimento nel Paese: hanno ottenuto meno risultati, perché non c'è stata nessuna operazione di regolarizzazione così generosa come in Italia; però hanno avuto la certezza di un reinvestimento nell'economia nazionale. Viceversa,

si può agevolmente vedere che sono tutti interventi di spesa corrente. Con un'entrata *una tantum* si finanzia spesa corrente. Si sarebbero potute fare scelte diverse; penso ad esempio al finanziamento di un piano per la mobilità nelle grandi aree urbane (abbiamo detto che ci condiziona fortemente la possibilità di raggiungere risultati in termini di clima); avremmo potuto investire sulla banda larga (una strozzatura dello sviluppo italiano); oppure sul fisco

il secondo elemento di giudizio è quello della rapidità dell'intervento. Ci sarebbero qui molte cose da dire ma non ho il tempo per farlo. Cito solo un elemento.

significa che nel cuore della più grave crisi degli ultimi 15 anni giacevano nel bilancio dello Stato 3,6 miliardi di euro inutilizzati; da almeno un anno erano lì e invece di essere impegnati

dell'Umbria, la regione che ho l'onore qui di rappresentare elettoralmente. Si tratta di una Regione, come voi sapete, ancora alle prese con la coda della ricostruzione del devastante terremoto che l'ha colpita, con le Marche, ormai 12 anni fa. Quindi, quella ricostruzione non è ancora terminata ed ecco, appunto, che un nuovo evento sismico colpisce una zona abbastanza estesa dell'Umbria, che si estende da porzioni del territorio di Perugia, tocca soprattutto i Comuni di Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e lambisce Todi. Quindi, è una zona abbastanza ampia. Mentre le prime notizie sembravano far profilare danni cospicui ma non devastanti, invece gli accertamenti stanno mettendo in luce un danno notevolissimo al patrimonio edilizio

che il sottosegretario Bertolaso, con la consueta solerzia e prontezza, si è già portato sul posto e ha compiuto una prima ricognizione. Debbo anche dire che la struttura della Protezione civile italiana (che ha già dato buona prova di sé in occasione degli eventi altrettanto gravi, o ancor più gravi, come quello abruzzese) ha risposto all'appello, alle esigenze dell'emergenza, talché i primi soccorsi sembrano essere stati apprestati con un'efficienza da sottolineare. voi comprendete bene che siamo in presenza, comunque, di un'emergenza, tanto più aggravata dalle inclementi condizioni del tempo che tanto bene, proprio in queste circostanze, si sono abbattute in generale su tutto il Centro Italia ma, in particolare, in queste zone terremotate. zone terremotate. Quindi, oltre naturalmente ad essere certo che questa Presidenza e l'intera Assemblea di Palazzo Madama vogliano indirizzare di tutto cuore ai miei concittadini dell'Umbria, così duramente provati, una manifestazione forte e unita di solidarietà,

riferisca a questa Assemblea, anche per rendere consapevoli gli onorevoli senatori in relazione agli interventi che si dovranno compiere e a